osservando, quanto all'articolo 9, l'opportunità che, in sede di emanazione dei decreti legislativi finalizzati alla individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sia assicurato il rispetto delle competenze regionali, individuando adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni. Si segnala inoltre, quanto all'articolo 12-*ter*, l'esigenza di assicurare il rispetto delle competenze regionali in materia di turismo. Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - sull'emendamento 26.0.800, parere non ostativo, a condizione che sia riformulato con la previsione dell'espressione del parere da parte della Regione interessata; - sui restanti emendamenti, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sulla proposta 26.0.551 (testo 2) parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - che alla lettera a), capoverso a-*bis*), dopo le parole "procedure selettive di cui alla lettera siano inserite le seguenti: "e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo,"; - che alla lettera b) le parole "valutati in " siano sostituite dalle seguenti: "pari Esprime poi parere non ostativo si tutti gli ulteriori emendamenti fino all'articolo 26-*quater.* Resta sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 27 in poi».

che penso si debbano intendere, come evidenziava il Servizio Studi, come siti istituzionali su reti telematiche - né dal punto di vista sostanziale. Ci troviamo di fronte, infatti, ad una rubrica dell'articolo 22 che parla dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e, all'interno di tale previsione, si arriva a chiedere che non vi sia più l'obbligatorietà della pubblicazione sui giornali

la valutazione del risarcimento del danno per il fatto che non si erogano servizi in modalità digitale. Francamente mi sembra scarsamente comprensibile. Forse sarebbe opportuno ritirarlo, tuttavia, se il presentatore insiste, si può accogliere.

garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

Presidente, con riferimento alle questioni che abbiamo sollevato questa mattina circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, prendo atto che il Governo ha opportunamente ritirato tre o quattro proposte di modifica, che erano chiaramente inammissibili.

l'oggetto del provvedimento al nostro esame e con l'elenco delle materie indicate nella risoluzione di approvazione del DPEF? Assolutamente nulla; quindi, la sollecito a dichiarare inammissibili tali emendamenti. Senatore Legnini, alcuni sono già stati respinti in Commissione e altri sono stati presentati per affinità,

palesemente estranei all'oggetto del provvedimento e all'elenco delle materie contenute nel DPEF e nella risoluzione che lo ha approvato. Lei dica se ciò che io ho contestato è vero o meno, perché se si limita a dire che invece queste materie sono trattate nel provvedimento

È fin troppo ovvio - e peraltro il nostro Regolamento, ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 126, lo stabilisce con solare chiarezza - che quando si esaminano disegni di legge collegati alla finanziaria, il vaglio sulla proprietà delle materie disciplinate dai testi, e dagli emendamenti addirittura, è assai più rigoroso di quanto non accada normalmente. Tanto è vero che la Camera o il Senato, a seconda di quale sia il ramo del Parlamento nel quale viene depositato depositato ed esaminato in prima lettura il disegno di legge collegato alla finanziaria, esegue un primo vaglio circa la congruità delle materie contenute rispetto ai documenti economici e un secondo vaglio, molto rigoroso, sugli emendamenti. Ora, in questo caso, ci stiamo stiamo trovando ad esaminare materie (rifiuti, acqua, incarichi dirigenziali, Consiglio di giustizia amministrativa) che non hanno relazione alcuna, non dico testuale, ma neanche di lontana affinità di materia, con il contenuto dei documenti economici. Presidente, questo è un tema molto serio, perché qui peraltro - me lo lasci dire - si gioca anche l'eguale opportunità dei giocatori di contribuire all'elaborazione di un testo, e possono passare, attraverso le dichiarazioni di ammissibilità e di inammissibilità, non solo strappi alle nostre regole, ma anche disuguaglianze rispetto al prodotto finale, ossia al provvedimento legislativo che questa Camera si trova ad approvare. Si tratta dunque di una questione molto delicata; non è una decisione che appartiene, come regolarmente accade, alla Presidenza in ordine al vaglio di qualunque emendamento presentato rispetto a qualunque provvedimento, per quanto regolato minuziosamente. Quello in questione è uno spazio regolatissimo, nel quale la discrezionalità, sostanzialmente non esiste, perché delle due l'una: o è materia riferita a parti e a disposizioni contenute nei documenti economici oppure non lo è, e in questo caso le suddette materie non lo sono.

*(PD)*. Signora Presidente, mi scuso, ma vorrei insistere sul punto sollevato dalla senatrice Finocchiaro e, prima ancora, dal senatore Legnini. La questione che riguarda il contenuto proprio dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria è regolata, con assoluta puntualità, dai nostri Regolamenti e dalla legge di contabilità, in modo tale che, alla fine, venga affidata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato, nel corso dell'esame di tali provvedimenti, la possibilità di pronunciarsi, preliminarmente e nel corso dell'esame, con assoluta sistematicità, sul carattere omogeneo al contenuto definito nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria di ogni provvedimento collegato non solo rispetto al suo titolo, ma, insisto, rispetto ai contenuti definiti

Se il Presidente della Commissione di merito li ha ammessi, ha valutato in modo che, a mio giudizio, non è corrispondente al nostro Regolamento, ma qui a decidere non è il Presidente della Commissione che ha esaminato il provvedimento, ma lei, cioè il Presidente del Senato. Quindi, la invito a riflettere sul punto su cui stiamo decidendo, perché cosa viene fuori se si continua con l'orientamento che lei ha già manifestato?

come tali proprio al fine di garantire che siano provvedimenti omogenei per materia. Ed è per questa ragione che si dice che bisogna fissarne il contenuto nella risoluzione Se poi invece la Presidenza del Senato, come in questo caso, ammette, violando palesemente il Regolamento e ciò che è previsto dalla legge di contabilità, che il provvedimento collegato possa, a sua volta, essere un provvedimento *omnibus* - e questo lo diventa se si dichiarano ammissibili emendamenti come questi - noi non solo non abbiamo semplificato la decisione di bilancio, ma abbiamo irrimediabilmente confuso, reso irriconoscibile, tutto il nostro procedimento legislativo. Mi spiace, ma si tratta di una questione delicatissima, su cui l'orientamento che sta prendendo la Presidenza mi pare lesivo gravemente del Regolamento e della legge di contabilità.

può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea».

ma soprattutto qui stiamo parlando di un testo in cui, durante il passaggio alla Camera, dove nasce a seguito di uno stralcio, è stato introdotto il tema del processo civile.

il pelo nell'uovo, potremmo aver fatto venti provvedimenti diversi per venti articoli, ma non credo che questo sia ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Oggi c'è bisogno di misure che favoriscano lo sviluppo economico e la semplificazione di di molti passaggi legislativi amministrativi, sia per la pubblica amministrazione sia per i privati. Io credo che questo prevalga di gran lunga rispetto ad ad un'aspirazione utopica di purismo della legislazione che, peraltro, non è mai stata attuata. Non parliamo certamente di questa legislatura, che è tutto sommato ai primi mesi, ma, se guardiamo Senatrice Finocchiaro, io non se ne avrà a male se dico che invocare la categoria del purismo è quanto meno incongruo rispetto a questo provvedimento e alla congerie di norme che contiene. Innanzitutto, lei ricorda male, collega: la questione che riguarda il processo civile stava nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria. questa materia la possiamo escludere dal novero. Così come assai difficilmente riesco ad introdurre, nelle norme che riguardano più complessivamente, come lei ha enunciato, il riordino dell'agire della pubblica amministrazione, le questioni relative agli incarichi dirigenziali. la spiegazione che ci ha appena fornito la Presidente dell'Assemblea dovrebbe tagliare il nodo gordiano di fronte al quale ci troviamo perché, al di là di ogni discussione che sta intercorrendo tra di noi sulla coerenza o meno delle materie qui

esso prevede che qualora fosse accaduto, contravvenendo alle regole precisamente enunciate nei commi 2-*bis* e 2-*ter*, che in Commissione si fossero introdotte norme, sia pure su emendamento, tali da proporre all'Assemblea un testo non coerente con l'elencazione delle materie della risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, in questo caso lei in questo caso lei avrebbe il dovere, come ha detto il senatore Morando, di espungere quelle parti e di dichiarare inammissibile ogni emendamento che tendesse a reintrodurle. È il terzo filtro, signora Presidente.

così è! E le dico anche, Presidente, che, poiché stiamo discutendo di una materia molto delicata che, come le ho detto prima, non riguarda soltanto l'osservanza delle regole che governano i nostri lavori, ma anche l'accesso, per una o per l'altra delle parti che stanno in questa Assemblea, Assemblea, alla possibilità di introdurre norme che le interessano in un testo, allora le dico che il mio Gruppo non è nelle condizioni di transigere su questo. Senatrice Finocchiaro, io riferirò al Presidente del Senato il senso delle sue osservazioni, ma, allo stato, non posso che ribadire le valutazioni della Presidenza già comunicate in mattinata circa l'ammissibilità degli emendamenti.

non mi sembrerebbe il caso di turbare il clima positivo che finora si era costruito su questo provvedimento (che, ricordo, è comunque un provvedimento collegato), per dare modo di riflettere e di calmare gli animi, sia opportuno, per il momento, accantonare gli emendamenti governativi aggiuntivi, riservandoci di valutarli e votarli nella prossima seduta. *(Applausi dal

nostri colleghi, i senatori Malan e Saro, sarebbero stati sostituiti nella Commissione affari costituzionali in quanto - sempre secondo quanto riferisce l'ANSA - dichiaratamente contrari al disegno di legge Calabrò.

Presidente, la prego vivamente di accantonare gli articoli 26-*bis*, che reca disposizioni concernenti la Corte dei conti,

Signora Presidente, non credo sia condivisibile la proposta del senatore Legnini di accantonare articoli che rientrano in un testo già approvato dalle Commissioni

una contiguità o addirittura una coincidenza di materia: nel momento in cui si predispone in un collegato la normativa relativa alla revisione del processo civile, il processo amministrativo, sostanzialmente, è materia analoga, in quanto disciplina disciplina forse non diritti, ma interessi legittimi che comunque attengono ai diritti delle persone all'andamento dei traffici. Perché nel collegato era stata inserita la riforma del processo civile? È ovvio: perché dalla giustizia civile dipende molto anche il grado di affidabilità, soprattutto internazionale, e di concorrenza di un Paese rispetto ai Paesi terzi. La stessa cosa vale per il processo amministrativo; poco si spiegherebbe perché, per avere giustizia in un'aula di tribunale civile, ci devono essere dei problemi e quindi va cambiata la procedura per incentivare gli investimenti nel nostro Paese, mentre sull'amministrazione, il cosiddetto *red tape*, rappresenta la parte più dolente, se vogliamo, dei motivi principali per cui sono più difficili gli investimenti esteri da noi, non tanto per il livello di tassazione, ma proprio per il livello di difficoltà che gli operatori hanno nei rapporti con l'amministrazione, non si vede dunque perché non si dovrebbe intervenire là La contiguità o similitudine di materia è talmente viva da far concludere che sostanzialmente tutta la materia processuale deve essere lavorata e riformata nell'ambito di questo provvedimento collegato. ho dimostrato la disponibilità del Governo ad accantonare gli altri emendamenti che introducono materie aggiuntive e sulle quali è opportuna una riflessione, su questi temi, che sono stati già ampiamente discussi dalle Commissioni riunite, francamente il Governo insiste per avere la votazione da parte del Senato.

mi dispiace non essere assolutamente d'accordo, sul piano rigorosamente regolamentare, con il sottosegretario Vegas. Infatti, la risoluzione la risoluzione di approvazione del DPEF parla esclusivamente di riforma del processo civile; il processo amministrativo è regolato da un'altra legge, riguarda un'altra giurisdizione e non ha nulla a che vedere con il processo civile. a cui si riferiva il sottosegretario Vegas, potremmo introdurre in questa legge il processo penale, il processo contabile, il processo del lavoro, il processo

non voler accantonare questi tre articoli che, oggettivamente, pongono problemi molto seri. Non capisco come si possa sostenere che la disciplina dell'Avvocatura dello Stato piuttosto che la materia pensionistica devoluta davanti alla Corte dei conti e quant'altro

Senatore Legnini, in assenza dell'unanimità dell'Aula, non possiamo che continuare i nostri lavori fino alle ore 19, come già annunciato dal presidente Schifani. Anche in questo caso, devo ribadire

seconda lettura, il Regolamento non ci consente di prendere in esame la questione di ammissibilità che, comunque, sottoponiamo alla Presidenza del Senato. Per questo motivo, non era compito della Commissione bilancio

Presidente, facciamo presente ai colleghi - non so dove sia ora la presidente Finocchiaro, ma spero che abbia la compiacenza di ascoltare - che si chiede lo stralcio di una norma introdotta dalla Camera dei deputati. Pertanto, non vedo come potremmo giudicare inammissibile una norma che nell'altro ramo del Parlamento è stata legittimamente varata e approvata. Non voglio fare il professore, ma credo che se questa fosse una sede d'esame, chi ha pronunciato quegli interventi verrebbe ampiamente bocciato. Ciò premesso, siccome un voto in più o in meno non cambia niente, noi rinunciamo a questa votazione, la faremo martedì, così la presidente Finocchiaro capirà che ha sostenuto una tesi sbagliata e che non ha subito, da parte nostra, alcuna prepotenza.

ad articoli approvati nelle Commissioni di questo ramo del Parlamento. Quindi, non dica cose non vere e non si riferisca in modo così irridente alla Presidente del nostro Gruppo. Ritiri quello che ha detto.

un minimo di tranquillità d'animo debba essere riportata in un dibattito che altrimenti rischia di andare fuori dai percorsi dell'ordinaria dialettica parlamentare e non se ne capiscono assolutamente i motivi, perchè fino ad ora abbiamo lavorato proficuamente su un testo che è indubbiamente complesso, ma che che tutto sommato mantiene un'unità logica indiscutibile. nello spirito di massima disponibilità per dare alla Presidenza, che è l'organo preposto alla decisione sull'ammissibilità degli emendamenti, un ulteriore tempo, se lo desidera, per valutare gli emendamenti stessi...

dichiarare inammissibili parti, o stralciare parti, accertando se ciascuna di esse «rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente» - e non è questa la fattispecie «nonché dal Documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare». Mi permetto, pertanto, di offrire alla valutazione della Presidenza le considerazioni che già avevo avanzato prima, vale a dire

di altre parti civili o della pubblica amministrazione, è di per sé inscindibilmente legata a quella del processo amministrativo. Questo è il punto sostanziale, per cui posso capire le contestazioni quando ci si riferisce al codice di dal senatore Legnini, che è tutt'altra cosa rispetto alle procedure civili. Oserei dire che anche il processo contabile è strettamente collegato alla procedura civile, perché verte sull'affidabilità e sull'affidamento dei diritti patrimoniali degli individui. individui. Questo, a mio sommesso avviso, è il punto. Quindi, non esiste un problema di incompatibilità di questa parte aggiunta dalle Commissioni rispetto alla finalità contenuta tra i collegati, come individuata dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Mi permetto semplicemente di offrire queste considerazioni alla Presidenza, affinché

valutare positivamente queste norme approvate dalla Commissione, il Governo - ovviamente deciderà l'Assemblea - non è sfavorevole a proseguire e a concludere questa parte del disegno di legge al più presto possibile, anche in questa seduta.